La seduta è aperta

Comunico che il Presidente del Senato, in data 17 maggio 2023, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, i senatori: Cantalamessa, Castiello, Della Porta, Aurora Floridia, Iannone, Melchiorre, Minasi, Mirabelli, Musolino, Nave, Paita, Potenti, Rando, Rastrelli, Russo, Sallemi, Salvitti, Scarpinato, Sigismondi, Silvestro, Sisler, Spelgatti, Ternullo, Valente e Verini. Il Presidente della Camera dei deputati, nella stessa data, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati: Antoniozzi, Ascari, Barbagallo, Bicchielli, Cafiero De Raho, Carrà, Castiglione, Colosimo, Congedo, D'Attis, De Corato, Gallo, Gubitosa, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Orlando, Piccolotti, Pittalis, Pretto, Provenzano, Serracchiani, Sudano, Tenerini e Zinzi. D'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione è convocata per procedere alla sua costituzione martedì 23 maggio 2023, alle ore 13, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo le senatrici Petrucci e La Marca. Comunico altresì che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima delegazione il deputato Centemero.

che il riconoscimento del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, dopo le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, impone allo Stato di porre in essere misure concrete in termini di interventi e risorse, al fine di riequilibrare, ovvero di ridurre, gli svantaggi economici e socioculturali derivanti dall'insularità, in attuazione altresì del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Gli interroganti richiamano anche i principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti regionali e locali e di sistema perequativo nella distribuzione delle risorse, ricordando come la legge delega di attuazione 5 maggio 2009, n. 42, sul cosiddetto federalismo fiscale e i relativi decreti legislativi non abbiano sortito i risultati attesi dal punto di vista della realizzazione di un efficace sistema perequativo a causa - si dice nell'interrogazione della mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard*. Secondo gli interroganti, le politiche pubbliche di intervento verso le aree insulari sono state assai poco efficaci in questi ultimi anni, al punto che è stato necessario l'intervento del legislatore costituzionale al fine di riconoscere la peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Con tali premesse, gli interroganti pongono il quesito in ordine alle iniziative del Governo e in particolare di chi vi parla, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per l'attuazione del principio costituzionale di insularità non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto i profili socioculturali. Orbene, non c'è dubbio che il riconoscimento costituzionale delle peculiarità delle isole sottende una valorizzazione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori e che la collocazione del più ampio principio di insularità all'interno dell'articolo 119 della Costituzione sia assai significativo. Com'è noto, l'articolo 119, dopo le modifiche introdotte con legge costituzionale n. 3 del 2001, ha inserito il principio del federalismo fiscale in Costituzione, recando la disciplina dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali corredata da un duplice sistema perequativo: un primo senza vincolo di destinazione in favore degli enti territoriali, con minore capacità fiscale per abitante, che è stato interpretato in sede attuativa come riferito a supportare le funzioni ordinarie degli enti territoriali (articolo 119, terzo comma); un secondo fondo di carattere strutturale per scopi diversi rispetto all'esercizio normale delle funzioni, ovvero la rimozione degli squilibri economici e sociali e l'esercizio effettivo dei diritti della persona (articolo 119, La previsione di un fondo perequativo, assente nel testo costituzionale previgente, che però prevedeva interventi statali a favore delle zone svantaggiate e delle isole è coerente con la logica complessiva del decentramento fiscale, in cui i territori sono responsabilizzati nelle scelte di spesa e nelle decisioni relative al loro finanziamento, in modo che ne possano rispondere ai propri elettori. In questo quadro, in sede di attuazione dell'articolo 119, dapprima con la legge delega n. 42 del 2009, di cui sono stato il principale promotore, e poi con i decreti legislativi attuativi, si è recuperato a vario titolo il riferimento all'insularità, al fine di assicurare interventi mirati a contrastare lo svantaggio naturale dei territori insulari e garantire un'effettiva parità con i cittadini della terraferma nel godimento dei diritti individuali e inalienabili. In particolare, la legge delega n. 42 del 2009 prevede all'articolo 22 disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale. Tale disciplina, oggetto di recente novella nel decreto-legge n. 121 del 2021, indica la specificità insulare tra le priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione. Il riconoscimento dell'esigenza di un intervento pubblico in relazione ai disagi connessi all'insularità è contenuto anche in interventi legislativi successivi alla legge n. 42, che sono diretti a specifiche realtà insulari - Sicilia e Sardegna - e non al complesso dei territori insulari. Alcuni interventi normativi hanno disposto finanziamenti *ad hoc* al fine di assicurare la continuità territoriale. Con particolare riferimento alle isole minori, che rientrano specificatamente nell'ambito della delega di funzione a me attribuita, in ordine al miglioramento delle prestazioni e all'efficacia della *governance* nei territori isolani, le isole presentano situazioni di svantaggio che riguardano vari ambiti: trasporti, ambiente, ridotta attività economica, scarsità di lavoro e problema demografico. Negli anni, lo sviluppo delle isole minori è stato anche sostenuto attraverso misure finanziarie specifiche, che hanno consentito investimenti importanti nei Comuni isolani. Un impatto significativo ha avuto anche l'introduzione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), un progetto volto a superare i differenziali negativi sottesi all'insularità rispetto a tre servizi essenziali per i cittadini: mobilità, istruzione e salute. Con il lancio della SNAI le isole minori sono state incluse nella progettualità delle amministrazioni centrali, con l'obiettivo di rendere le isole minori una sorta di 73a area interna, a fronte delle prime 72 già finanziate, destinatarie di risorse e interventi volti a favorire lo sviluppo locale e il contemperamento di distanza e isolamento nell'offerta dei tre citati servizi di cittadinanza. In questo quadro, la mia azione di Governo si sta muovendo su un duplice binario a favore dei territori insulari. Da un lato, la valorizzazione delle isole si colloca nell'ambito del processo di attuazione dell'autonomia differenziata prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Com'è noto, il mio disegno di legge sull'autonomia differenziata, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionale del Senato, contiene uno specifico riferimento ai territori insulari, laddove prevede (all'articolo 9) misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. Contestualmente sarà fondamentale, per i territori insulari, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP), ad opera della cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023 e supportata da un apposito comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il compimento del processo di definizione dei LEP, dei fabbisogni e dei costi *standard*, determinando l'ammontare del servizio o della prestazione che deve essere garantito dal settore pubblico in modo uniforme sul territorio e quindi anche sui territori isolani, costituisce un lavoro imponente che può portare a una piena attuazione dell'articolo 119 e a una perequazione effettiva nei territori svantaggiati come le isole. Parallelamente, lungo un'altra direttrice, il tema delle isole minori rappresenta una priorità per la mia azione di Governo. A tal fine, anche attraverso il dialogo con le amministrazioni locali dei territori isolani e con le associazioni di categoria, sto mettendo a punto un disegno di legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, volto a superare la frammentazione normativa che finora ha caratterizzato le iniziative a favore di queste ultime. Il disegno di legge che mi appresto a presentare in Consiglio dei ministri indica misure di crescita per le isole minori (marine, lagunari e lacustri), in considerazione del loro valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate. Esso reca disposizioni in linea con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla tutela delle aree insulari, attraverso provvedimenti e normative specifici per superare i divari geografici, infrastrutturali amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari. Il testo che si intende presentare al Parlamento, prendendo spunto dalle disposizioni contenute nel disegno di legge di iniziativa parlamentare approvato in prima lettura al Senato all'inizio della scorsa legislatura e che si era arenato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene, rispetto a quest'ultimo, modifiche sostanziali al fine di migliorarne la coerenza organica e la portata applicativa. Innanzi tutto, interviene sulle risorse a favore delle isole minori, incrementando il fondo di sviluppo delle isole minori e istituendo un nuovo fondo di sostegno per gli investimenti nelle isole minori. Prevede poi la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tipicità delle isole minori e interviene sul tema dei servizi pubblici attraverso misure volte a migliorare, a vario titolo, l'assistenza sanitaria e la continuità del sistema scolastico nelle isole minori. Anche in materia di trasporti, l'obiettivo dell'intervento va nel senso di garantire nelle isole minori la continuità territoriale con la terraferma, al fine di migliorare tutti i tipi di collegamento. Sono previste forme di collaborazione con università e istituti di ricerca per favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori e accordi con istituti di credito per incentivare il tessuto produttivo locale e lo sviluppo del lavoro che non può essere solo stagionale - nonché norme a tutela dell'ambiente nelle isole minori. Si fa riferimento in particolare alla gestione dei rifiuti, alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, alla facoltà per le Regioni territorialmente competenti di predisporre un piano per promuovere la desalinizzazione delle acque nonché la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. conclusione, l'obiettivo è definire una legislazione quadro che, per lo sviluppo delle isole minori, agevoli le politiche di intervento pubblico in settori diversi e in una prospettiva non esclusivamente economica, ma anche culturale e sociale. Signor Presidente, saluto e ringrazio il signor Ministro per la risposta all'interrogazione che ho presentato il 27 dicembre scorso.

e c'è parecchia discordanza. Ha annunciato la legge quadro e ovviamente la aspettiamo; vigileremo sulla sua applicazione e sulla sua attuazione. Parliamo però di oggi: il principio di insularità non può essere nascosto - questo l'ho rimarcato nella mia interrogazione e nella sua risposta lo ha fatto anche lei - o addirittura schiacciato dall'aspetto economico-finanziario, perché così non risolviamo nulla. L'insularità è una condizione geografica i cui riflessi economico-finanziari rappresentano una delle tante conseguenze, al pari delle ricadute sociali, umane, culturali e storiche che ne derivano. Il principio di insularità chiede il rispetto, ancor prima che dell'articolo 119 della Costituzione, dell'articolo 3, che sancisce un principio di uguaglianza formale, ma soprattutto sostanziale. Auspichiamo quindi che questa maggioranza si focalizzi sulle vere necessità dei territori insulari e non sull'approvazione di un disegno di legge di autonomia finanziaria, che - mi scusi, signor Ministro - per le isole non fa nulla. Lei ha parlato di riferimenti, ma non è assolutamente sufficiente. Sarebbe auspicabile partire dalla previsione di un sistema di trasporto efficace ed efficiente, e non dalla creazione di ulteriori disuguaglianze tra le Regioni. La distanza geografica delle isole si trasformerà, anzi si sta già trasformando in una vera e propria distanza sociale. Nel caso della mia Regione, signor Ministro, è difficile per un sardo sentirsi parte integrante della Repubblica quando si ha il coefficiente di infrastrutturazione più basso della Nazione, quando Nuoro è l'unico capoluogo di provincia in Italia a non essere servito dalla rete ferroviaria nazionale o quando si si deve sperare che non ci siano scioperi dei voli per poter tornare a casa. Signor Ministro, siamo veramente preoccupati, perché il vostro disegno di legge rafforza queste disuguaglianze e a certificarlo è stato il Servizio del Bilancio; altro che principio di insularità. Mi perdoni, signor Ministro, ma ancora una volta è venuto meno il senso istituzionale. I funzionari del Senato hanno sollevato questioni di merito sul disegno di legge per l'autonomia differenziata; il Servizio del Bilancio ha posto una questione tecnica, non politica. Come si pensa di conciliare la concessione di nuove funzioni differenziate alle Regioni senza pregiudicare il godimento dei LEP nelle altre Regioni, il tutto in totale invarianza finanziaria? Per questo i funzionari sono stati richiamati? Altrimenti, come dobbiamo interpretare la modifica del *dossier* avvenuta con l'inserimento di un sottotitolo insolito: «Bozza provvisoria non verificata»? Ci chiediamo, a questo punto, chi dovrebbe verificarla; non la sua segreteria politica. Anzi, lo chiedo: la sua segreteria politica? Chi? Sono insoddisfatta della sua risposta e sono preoccupata per quanto è successo e per quello che potrebbe succedere. Emerge in tutto questo una differenza profonda tra due modi di lavorare, a nostro avviso: da questa parte, si chiede e si lavora per ridurre le disuguaglianze; voi, signor Ministro - mi dispiace - per aumentarle.

Signor Presidente, signori senatori, l'interrogazione muove da una notizia pubblicata dalla testata giornalistica «Il Riformista», secondo la quale la Romeo Gestioni SpA, società aggiudicatrice dell'appalto indetto da Adisurc per la gestione di residenze universitarie, si è vista esclusa dall'aggiudicazione per aver inserito all'interno del servizio di portierato lavoratori con disabilità, senza che il ricorso a tali figure fosse stato riportato dal progetto tecnico in sede di presentazione dell'offerta. A seguito delle verifiche effettuate dai miei uffici, abbiamo appurato che l'esclusione è stata oggetto di impugnazione da parte della Romeo Gestioni SpA innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, registrata come atto 177/2013 e che uno dei punti di censura verte sulla mancanza dell'idonea rappresentazione del modello organizzativo al momento dell'offerta. Pertanto, la vicenda è al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza tenutasi proprio lo scorso 9 maggio. È del tutto evidente, dunque, che non posso pronunciarmi sulla questione specifica dovendo la magistratura ancora accertare In termini generali, la tematica relativa all'impiego di lavoratori con disabilità, come disciplinata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, esula dalle mie strette competenze. Aggiungo quindi solo una puntualizzazione fornita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La legge n. 68 del 1999, all'articolo 3, prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, ossia persone in età lavorativa con disabilità fisica, psichica o intellettiva nella seguente misura: dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

due precisazioni che riguardano davvero l'inclusione lavorativa. Innanzitutto, mi auguro che tutte le aziende del nostro Paese adempiano a quanto prescritto dalla legge n. 68, e non solo perché è un obbligo, ma perché tutte le persone hanno diritto a essere valorizzate e inserite nel mondo del lavoro. Detto ciò, mi auguro anche che che tutte le aziende valorizzino tali competenze allo stesso modo di quelle di tutti gli altri lavoratori, quindi con una retribuzione equa e davvero davvero di pari opportunità per tutti i lavoratori con disabilità. Sicuramente la legge n. 68 ha bisogno di essere riformata, attualizzata, riadeguata, ma credo che serva davvero anche un grande salto di qualità del nostro Paese, un cambio di prospettiva: da quello di doversi attenere ai meri obblighi di legge da quello di doversi attenere ai meri obblighi di legge a quello invece di valorizzare le competenze in tutte le persone, soprattutto in quelle più fragili, che hanno bisogno non solo di essere aiutate, ma anche di avere un'occasione e una possibilità per poter lavorare nel nostro Paese

Lei non ha risposto entrando nel merito dell'articolo 4 della Costituzione, che voglio ricordare: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo Nello specifico, la sua risposta non fa chiarezza sulla natura discriminatoria delle clausole di questo appalto che, di fatto, hanno impedito a persone con disabilità - e qui cito la parte seconda dell'articolo 4 della Costituzione «di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Noi dobbiamo investire nel talento e nelle competenze di tutti, ma ancor di più delle persone con disabilità, garantendo realmente l'accessibilità fisica agli spazi e ai servizi nel pubblico e nel privato. Con il primo dei decreti attuativi della legge delega sulla disabilità, di recente approvato, ci auguriamo che almeno le amministrazioni pubbliche si adeguino velocemente. Sappiamo che, entro la primavera del 2024, gli altri quattro decreti dovranno essere attuati e noi vigileremo, come forza di opposizione, su di essi.

bisognava rispondere anche sul diritto al lavoro, sulla ferita che è stata inferta da un ente pubblico che praticamente ha negato l'accesso al lavoro a dei disabili.

Grazie,

che favoriscono l'inserimento lavorativo a giovani con disabilità - questo glielo ricordo io - se si è impotenti contro una Regione che mette alla porta persone con disabilità che vogliono lavorare.

Quindi, io credo che il lavoro per i disabili sia un'emergenza vera, una priorità vera, anche perché produrre reddito significa strappare alla povertà le persone con disabilità e le loro famiglie. Anche questo, però, mi sembra che non sia stato fatto nel recente decreto lavoro. Mi dispiace dirlo, ma le destre hanno totalmente relegato in un angolo il tema della disabilità, denunziato da diverse associazioni di categoria. A tal proposito, faccio mia la posizione del Coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di Down, che ha letteralmente bocciato le disposizioni in materia di disabilità contenute nel decreto. Allo stesso modo, la disciplina prevista per l'assegno di inclusione prevede parametri così stringenti che, di fatto, escluderà cittadini portatori di disabilità che versano in condizioni economiche critiche. Il rischio è che un adulto solo, cui è riconosciuta l'indennità di accompagnamento oltre alla pensione, ma con ISEE pari a zero, non potrà accedere all'assegno di inclusione. Mi scusi, ma questa è una vergogna, parlando proprio di inclusione. non spetta certamente a me ricordare come l'approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che il signor Ministro conosce bene, è un importantissimo traguardo, che le leggi italiane

chi rischia di rimanere indietro, in particolare i cittadini portatori di disabilità, che chiedono non privilegi, ma solamente il rispetto dei propri sacrosanti diritti.

Signor Presidente, riguardo le questioni poste, si specifica quanto segue. Innanzi tutto, si deve precisare che i valori limite previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 trovano fondamento nell'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria. Pertanto, un'eventuale fissazione e un'imposizione di nuovi valori limite di determinate sostanze dovrebbero scaturire da approfondite analisi e valutazioni che tengano in conto le ricadute sanitarie, così come i costi e la fattibilità tecnica nel raggiungimento di nuovi valori soglia. Si evidenzia come la stessa OMS indichi che i valori inseriti nello studio del 2021 rappresentano quelli a cui tendere nel medio periodo, e pertanto non da raggiungere nell'immediato. Peraltro, dallo scorso ottobre è in corso il negoziato presso il Consiglio del Parlamento europeo della nuova direttiva sulla qualità dell'aria, in cui verranno definiti i nuovi valori limite con previsioni di fine lavori nel corso del 2024. Riguardo i grandi impianti industriali, oltre ai limiti di legge in termini di concentrazione, si applicano i principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento introdotti dall'ordinamento comunitario

strategici di interesse nazionale, fra cui lo stesso stabilimento, trova applicazione la legge n. 231 del 2012, che ha introdotto l'obbligo per tali impianti della redazione di un rapporto di valutazione del danno sanitario, applicando i criteri metodologici definiti dal decreto interministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero della salute. Nel caso specifico di Taranto, le valutazioni sanitarie sono elaborate annualmente ai sensi del citato decreto interministeriale dall'Agenzia regionale per la (ISPRA) invece conduce le attività di verifica del rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi correlati all'esercizio dello stabilimento siderurgico, secondo il piano di monitoraggio e controllo ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016. Il monitoraggio della qualità dell'aria viene condotto dall'ARPA Puglia attraverso la rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, conformemente ai criteri stabiliti dal menzionato decreto legislativo n. 155 del 2010. I dati, una volta validati, sono pubblicati sul sito dell'Agenzia. In particolare, nei comuni di Taranto e Statte sono presenti numerose stazioni di misurazione della qualità dell'aria. Inoltre, la prescrizione n. 85 del decreto del riesame dell'AIA n. 547 dell'ottobre 2012 ha prescritto l'installazione di sei stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria in prossimità del perimetro dello stabilimento. L'ISPRA stesso, a seguito delle criticità segnalate da ARPA Puglia e ASL Taranto del dicembre 2022, ha avviato una serie di attività finalizzate a ricercare fattori oggettivi che, all'interno dello stabilimento siderurgico e dei complessi industriali soggetti ad AIA nazionale e limitrofi, possono determinare l'incremento delle concentrazioni di benzene fino a livelli molto

con particolare riguardo alle relazioni fra emissioni, concentrazioni ambientali ed esposizione della popolazione, al fine di individuare le attività specifiche all'origine della criticità e di individuare misure idonee alla prevenzione del rischio. Per tale motivo, il controllo ordinario relativo al primo trimestre 2023 per lo stabilimento ADI è stato realizzato definendo, in collaborazione con ARPA Puglia, uno specifico piano di ispezione incentrato sugli impianti per i quali il benzene risulta essere un inquinante pertinente. Sono stati ricercati eventuali fattori di aumento di benzene anche nel corso della visita ispettiva ordinaria, condotta nel marzo scorso presso gli impianti ENI raffineria di Taranto ed ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso di realizzazione anche presso la centrale termoelettrica ADI Energia. Si evidenzia inoltre che, in relazione al monitoraggio di emissioni fuggitive, polveri, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzene provenienti dalle aree a caldo dello stabilimento, sono in fase di esecuzione da parte di ISPRA approfondimenti e valutazioni sui monitoraggi effettuati presso le centraline di qualità dell'aria ubicate all'interno dello stabilimento, che vengono analizzate da ARPA Puglia al fine di monitorare gli andamenti dei profili emissivi negli anni, con eventuali ipotesi di correlazioni alle sorgenti rispetto ai monitoraggi previsti dalle prescrizioni del piano di riesame. Dalle valutazioni in corso si evidenzia una significativa variabilità negli anni, mentre l'eventuale correlazione con le criticità segnalate nelle aree a caldo è oggetto di particolare approfondimento, al fine di poter proporre possibili misure mitigative o preventive da adottare, che potranno essere oggetto della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare, per il parametro benzene si osservano valori isolati, acquisiti su base settimanale secondo la prescrizione 30, sul piano di carica delle batterie, che superano alcune unità di milligrammi per metro cubo. Per tali criticità sono attualmente in corso ulteriori indagini mirate. Inoltre, ISPRA sta verificando e valutando, in collaborazione con ARPA Puglia, di eseguire accertamenti strumentali in specifiche aree dello stabilimento siderurgico, nonché in altre aree della limitrofa raffineria ENI, al fine di valutare la possibilità di posizionare specifici campionatori passivi per condurre monitoraggi continui in aggiunta alle centraline già esistenti, con lo scopo di valutare i contributi delle eventuali fonti da cui si originano i crescenti livelli di benzene, così come segnalato da ASL Taranto e ARPA. Anche a fronte di accertamenti di inosservanze nel corso degli anni, per cui è stata informata la prefettura di Taranto, si evidenzia di Taranto, si evidenzia un sostanziale bilanciamento tra gli esiti nell'applicazione della normativa speciale applicata al caso di Taranto. Studi predittivi sugli effetti sanitari, quali la valutazione di impatto sanitario (VIS), risulteranno certamente utili anche ove si configurassero significative modifiche all'assetto produttivo o al contesto ambientale e sanitario, anche in riferimento ai criteri metodologici per la redazione della VIS, predisposti dall'Istituto superiore di sanità nel 2019, anche in vista di un rinnovo del riesame dell'AIA. Pertanto, qualora l'istanza del rinnovo prospettasse assetti produttivi significativamente differenti da quelli in essere, sarà facoltà delle autorità sanitarie richiedere specifici approfondimenti per poter definire in proposito le proprie determinazioni.

per ritardi e inadempienze e in scadenza il prossimo 23 agosto; dall'altra, si chiedeva se era intenzione del Governo condizionare il rilascio della nuova AIA ad una nuova e preventiva valutazione dell'impatto ambientale e sanitario. Su questi due principali aspetti dell'interrogazione non si sono fornite risposte, dimostrando peraltro di non conoscere la complessa realtà dello stabilimento ex ex Ilva, tuttora sotto sequestro, su cui sono intervenute diverse sentenze, anche del tribunale di Taranto e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e su cui permane ancora un rischio di infrazione europea da oltre dieci anni. Per queste ragioni, riteniamo la risposta del Governo e dei Ministri interpellati assolutamente insoddisfacente. Proverò nel poco tempo a disposizione a sintetizzare le criticità e a fornire al Governo alcuni suggerimenti, che spero possa considerare nel corso del riesame dell'AIA. È bene innanzitutto considerare l'ultimo rapporto di valutazione del danno sanitario, pubblicato a giugno del 2021 dall'OMS, che conferma le precedenti valutazioni e attesta la permanenza di un residuo rischio cancerogeno inaccettabile, relativo all'attuale produzione autorizzata di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio. mondiale della sanità calcola sullo scenario produttivo pre-AIA 2010 addirittura un *range* di decessi prematuri evitabili tra i 270 e i 400 adulti *over* 30;

tra 50 e 80 unità, ma non si azzererebbero comunque. Lo studio peraltro non considera gli ulteriori effetti negativi, come i decessi dell'età infantile dei giovani *under* 30, dell'esposizione congiunta e prolungata ai diversi inquinanti, nonché l'inquinamento del suolo e delle acque. Allo stesso tempo, l'OMS ha stimato il danno economico, dovuto solo alla mortalità prematura degli *over* 30, rispettivamente nei periodi osservati, tra gli 85 e i 15 milioni di euro annui. Per queste ragioni, chiediamo al Governo di confermare la validità delle valutazioni del danno sanitario, così come attestate, in ultimo, dall'OMS; verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni AIA 2012, perché sarebbe assurdo concedere un'ulteriore proroga o una nuova AIA laddove non risultassero rispettate le prescrizioni della prima, ovvero condizionare il riesame della nuova AIA ad una nuova valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario, in modo da stabilire in maniera scientifica se l'impianto siderurgico di Taranto sia nelle condizioni di produrre senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e quali siano eventualmente i limiti produttivi accettabili. Inoltre, rappresentanti del Governo, avete avviato la consultazione pubblica per il riesame della nuova laddove il documento pubblicato presenta *file* secretati e non accessibili ai cittadini, contrariamente a quanto accaduto in passato e in evidente violazione dei principi di trasparenza. Infine, signori del Governo, sul piano sostanziale,

In particolare, il riesame dell'AIA prevede la riattivazione dell'altoforno 5, il rifacimento dell'altoforno 3, la riattivazione delle batterie 3 e 4 e persino la trasformazione dell'altoforno 2 in un vero e proprio inceneritore. Si prevede di bruciare persino materiale plastico, fino a 60.000 tonnellate annue. Tutto questo significa continuare ad autorizzare l'uso del carbone. Chiedo al Governo se sia questo il processo di decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva. Intendete sostenere la transizione ecologica? Vi do solo alcune indicazioni: nelle 32 pagine lette della sintesi non tecnica sapete quante volte il termine «carbone» è ripetuto? Ben 28 volte. Sapete quante volte

Si comprende bene quali sono gli orientamenti del Governo: continuare a produrre a carbone. Per questo motivo avete introdotto lo scudo penale, proprio per proteggere i responsabili dai reati penali. Signor Presidente, concludo. Abbiate il coraggio di venire a Taranto e di dire ai cittadini di Taranto e ai lavoratori che questo è il modello produttivo che state sostenendo e finanziando, peraltro con i 680 milioni di euro che avete regalato per questa attività produttiva. Su questo noi saremo contrari. Chiediamo invece al Governo un accordo di programma e un atto di coraggio, che preveda la chiusura delle fonti inquinanti e adeguate tutele a favore dei lavoratori, delle imprese dell'indotto e dell'intera comunità.

Signor Presidente, con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli interroganti avanzano quesiti specifici in ordine alla possibilità di ripristinare le disposizioni in materia di colloqui telefonici dei detenuti, adottata nel corso dell'emergenza pandemica, anche valutando una relativa messa a regime, alla luce delle ricadute avute nel corso degli ultimi due anni, ritenute positive. Orbene, in effetti, la disciplina emergenziale stilata nel periodo pandemico n. 34 del 2020), oggetto di più deroghe, è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2022 e prevedeva oggettivi ampliamenti in tema di colloqui telefonici tra detenuti e familiari.

che queste devono essere favorite poiché, oltre ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari, evitano altresì trasferte costose e insostenibili fisicamente per anziani e malati e psicologicamente stressanti per i figli minori, nonché rendono non necessarie le lunghe e defatiganti operazioni di perquisizione dei soggetti che fanno ingresso in istituto in occasione dei colloqui in presenza. Inoltre, le videochiamate, applicate inizialmente in via sperimentale ai soli detenuti del circuito media sicurezza, in base alle modalità dettate con precedentemente circolare DAP del 30 gennaio 2019, dovevano essere estese anche ai detenuti di alta sicurezza, tenuto conto degli effetti positivi che il loro ricorso ha comportato sul piano trattamentale. Quanto alle conversazioni telefoniche, invece, la citata circolare ha ben fornito indicazioni operative valide anche per il prossimo futuro, stabilendo che in linea generale le telefonate possono essere autorizzate anche una volta al giorno, ove riguardino figli minori e figli maggiorenni portatori di una disabilità grave, oppure il coniuge, l'altra parte dell'unione civile e una persona stabilmente convivente o legata da relazione stabilmente affettiva, il padre, la madre, il fratello e la sorella del condannato, qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Da tali indicazioni sono escluse le persone detenute o internate sottoposte al regime previsto dall'articolo 41*-bis* per le quali si applicano le prescrizioni dettate dalla normativa, ovvero il detenuto o internato può essere autorizzato a fruire di un colloquio telefonico mensile dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, in alternativa al colloquio visivo. invece previsto che, nel caso di soggetti non sottoposti a tale regime, ma comunque detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4*-bis* dell'ordinamento penitenziario*,* l'autorizzazione della comunicazione telefonica non sostitutiva del colloquio in presenza non può essere concessa più di una volta a settimana. In conclusione, già in attuazione della recentissima circolare soprarichiamata, le direzioni degli istituti, laddove ne venga a rilievo la competenza e compatibilmente con le esigenze organizzative delle singole strutture penitenziarie, accordano le autorizzazioni in maniera consapevolmente ampia, specie in presenza, oltre che per le situazioni già tipizzate dalla norma, anche in caso di difficoltà dei visitatori a raggiungere gli istituti in ragione delle distanze dal luogo di residenza o di concorrenti impegni lavorativi o familiari.

siamo abbastanza stupiti dal fatto che né il Ministro né alcuno dei tre Sottosegretari abbiano ritenuto opportuno e abbiano trovato il tempo di venire a rispondere su un'interrogazione che riguarda una questione così delicata come la condizione dei detenuti nei nostri penitenziari. Detto questo, sono

dei penitenziari di valutare come e quando consentire le chiamate telefoniche. Voglio ricordare che oggi la regola di base è che è consentita una chiamata settimanale ai detenuti per dieci minuti. Questa regola è stata derogata

Questa condizione è stata resa possibile da norme che sono state prorogate continuamente nel corso della pandemia e che poi, da ultimo, non sono state prorogate. Ora non possiamo accontentarci di dare ai direttori degli istituti penitenziari un'ampia discrezionalità nella scelta, perché questo crea una disparità di trattamento

che si può attuare con facilità, che è stato sperimentato, che non ha dato problemi, che è in linea con la progressività del trattamento penitenziario, per cui, laddove le norme di favore vengano attuate con attenzione con attenzione e non provochino problemi, è opportuno estenderne la validità. Penso che non ci possiamo accontentare della risposta che ci ha dato il Ministero, che non ci possiamo accontentare di questa situazione a a macchia d'olio, di discrezionalità lasciata ai direttori, ma che occorra intervenire normativamente per consolidare una condizione che si è attuata negli ultimi due anni, che ha dato buona prova e che è un grave errore non prorogare anche per il futuro.

energetica*. Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante, riferite le criticità di organico rilevabili nel carcere di Potenza, avanza quesiti sulle iniziative che si intendono perciò

riduzione, com'è noto, è stata operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista altresì da successivi interventi normativi che hanno rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del Corpo della polizia penitenziaria e su cui andrà evidentemente reimpostata una politica di implementazione. Sul punto, giova evidenziare che allo stato, a fronte di un organico totale di 42.150 unità, come dall'ultimo incremento di 1.000 unità del ruolo di agenti assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - il personale del Corpo di polizia penitenziaria amministrato ammonti a 36.126 unità. Va inoltre rammentato che, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al *turnover*, l'assunzione straordinaria di complessive 2.804 unità. Ciò precisato, sempre ai fini di razionalizzazione ed efficienza, nonché di adeguamento degli interventi legislativi *medio tempore* intervenuti, è in via di predisposizione il nuovo decreto ministeriale, che andrà a sostituire il decreto ministeriale 2 ottobre 2017, per la redistribuzione della dotazione organica del Corpo. Tornando alla carenza di personale in generale, si rappresenta che sono in essere varie procedure concorsuali, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste. Quanto alla carenza di commissari, è in essere il concorso pubblico per 120 posti, in relazione al quale si sono conclusi gli accertamenti psicofisici e attitudinali. È in essere poi il concorso pubblico per complessivi 411 allievi di vice ispettore, nonché quello per complessivi 1.758 allievi agenti. Dette procedure concorsuali saranno concluse entro il corrente anno. Inoltre, in data 15 marzo 2023, è stato pubblicato il nuovo concorso allievi agenti per 1.713 posti. Quanto alle procedure interne, merita rammentare il concorso per complessivi 691 posti di ispettore, la cui procedura si è conclusa, nonché il concorso per titoli a 583 posti, poi elevati a 813, di vice sovrintendente, l'inizio quali era datato al gennaio 2023. Infine, merita rammentare che è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti, che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e 361 unità del ruolo femminile. Quanto alla situazione del carcere di Potenza, si evidenzia che, a fronte di un organico previsto pari a 122 unità, ne risultano presenti 112, comprese sei distaccate in uscita e undici in entrata, inferiore dunque di dieci unità rispetto a quella prevista. Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo di sovrintendenti (meno sei unità) e degli agenti assistenti (meno dieci unità). Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si evidenzia che, in esito al concorso interno per complessivi 583 posti, il DAP ha già previsto di assegnare alla casa circondariale di Potenza quattro unità maschili e un'unità femminile, il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione. Quanto al ruolo di agenti assistenti, si rappresenta che l'organico dell'istituto di Potenza è stato incrementato, nell'anno 2022, di sei unità maschili e quattro unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 180° corso.

in cui si trovano le carceri e soprattutto le condizioni in cui si trova ad operare la Polizia penitenziaria. Quest'interrogazione nasceva anche dal fatto che a Potenza tra qualche mese, dopo mesi di ristrutturazione, riaprirà il settore femminile

una carenza di organico. Riaprirà inoltre il primo settore maschile, che era stato anch'esso chiuso per ristrutturazione. Io spero che, a seguito di tutte queste assunzioni e dei concorsi che sono stati previsti, il Ministero preveda un incremento delle unità presso il carcere di Potenza, perché questo significa una migliore qualità del servizio, una migliore qualità del lavoro da parte della Polizia penitenziaria e una maggiore sicurezza in concreto. Sono quindi fiducioso che, a seguito di questo impegno da parte del Governo a rimpinguare le Forze di polizia, ci sarà attenzione anche per l'istituto penitenziario A. Santoro di Potenza.

alle quali risponderanno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Signor Presidente, gentile Ministra, mi permetta di riassumere il contenuto della mia interrogazione, indirizzata al Ministero del lavoro, ma di grande interesse anche per il Ministero del turismo, per cui sono particolarmente contento della presenza anche della ministra Garnero Tutti i dati e le note previsionali, compresi quelli del Ministero del turismo, indicano un forte incremento della presenza turistica in Italia, con un effetto positivo dell'ordine di 89 miliardi di euro sulla spesa turistica, pari a un aumento del 22,8 per cento rispetto allo scorso anno. Con il DPCM del 29 dicembre 2022 il Governo ha autorizzato l'ingresso in Italia di 82.700 lavoratori stranieri, di cui 44.000 per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero e in quello agricolo e 38.000 per lavoro non stagionale e autonomo. Lo scorso 27 marzo, in occasione del *click day*, i datori di lavoro hanno formulato richieste per circa 250.000 lavoratori stagionali, evidenziando l'enorme differenza tra i flussi di ingresso regolari autorizzati e il fabbisogno necessario. Con la successiva attribuzione territoriale delle quote agli ispettorati territoriali, i datori di lavoro, in particolare quelli del settore alberghiero, hanno dovuto amaramente prendere atto della decurtazione delle quote. A fronte di una richiesta di circa 40.000 ingressi per l'anno 2023, di cui 30.000 stagionali e 9.250 non stagionali, gli ingressi per lavoro stagionale destinati al settore alberghiero sono stati decurtati a sole 20.500 unità. In particolare, nella sola provincia autonoma di Bolzano, a fronte della stima di un fabbisogno di forza lavoro di circa 600 quote per lavoro stagionale e 100 quote pluriennali, sono state assegnate unicamente 138 quote stagionali, 24 quote pluriennali pluriennali e 317 quote con riferimento alle organizzazioni professionali dei datori di lavoro. È evidente che tutto questo sta ingenerando enorme preoccupazione. Si chiede allora se, per venire incontro alle esigenze manifestate dai di lavoro, non si intenda integrare le quote previste, scongiurando così il rischio che un settore strategico come quello del turismo possa risentire nella qualità dell'offerta per mancanza di manodopera. Grazie, signora Ministra.

dicembre 2022 sulla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il 2022, sono stati definiti gli ingressi in Italia per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, e di lavoro autonomo di cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità, come si diceva, di cui 38.000 destinate a ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, in quello turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni e nei settori alimentare e della cantieristica navale, per lavoro autonomo e per le conversioni dei permessi di soggiorno, e 44.000 unità destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Con particolare riferimento all'oggetto del quesito, nell'ambito della quota complessiva di 44.000 unità, 1.500 sono riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale 22.000 quote sono riservate per il settore agricolo ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate in nome e per conto dei datori di lavoro dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro. Con nota del 30 marzo 2023, correttamente richiamata dai senatori, la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attribuito agli ispettorati territoriali del lavoro le quote per lavoro subordinato, di cui agli articoli 3, 4 e 6 del DPCM, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione. Con riferimento alle 44.000 quote di lavoro stagionale, sono state distribuite agli ispettorati generali del lavoro, Regioni e Province autonome tutte le quote previste dal decreto, proporzionalmente ed in base alle istanze presentate dai datori di lavoro e comunicate dal Ministero dell'interno lo scorso 28 marzo e non sulla base delle richieste formulate dalle amministrazioni. In particolare, il Ministero dell'interno ha riferito che alla data del 15 maggio risultano pervenute complessivamente 286.946 istanze, di cui 168.288 per lavoro stagionale. A seguito delle segnalazioni pervenute sull'insufficienza delle quote di ingresso assegnate per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori dell'agricoltura e turistico-alberghiero, nella consapevolezza della rilevanza degli interessi sottesi a questa richiesta, ossia la necessità di dare una risposta al sempre più crescente fabbisogno di manodopera in questi settori, il Ministero del lavoro ha posto in essere gli adempimenti necessari per l'assegnazione di quote aggiuntive di lavoro stagionale e pluriennale nei settori interessati. Con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, sono state assegnate ulteriori 359 quote, per un totale di 600 quote di lavoro stagionale e 100 quote di lavoro stagionale pluriennale, come da fabbisogno segnalato dalla commissione provinciale a gennaio 2023. Faccio presente, inoltre, che per il triennio 2023-2025, il decreto 20 marzo 2023, n. 20, ha previsto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il fatto di ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e autonomo, altre quote. Ecco perché

Ringrazio per l'assegnazione di queste quote aggiuntive, veramente sentite nel nostro territorio. Voglio rivolgerle anche un ringraziamento personale, per la sua disponibilità agli incontri anche con le nostre piccole realtà nella Provincia autonoma di Bolzano, per risolvere i problemi concreti che abbiamo.

premesso che nella scorsa legislatura è stato introdotto il cosiddetto reddito di cittadinanza, strumento che, nelle previsioni delle forze politiche promotrici, avrebbe dovuto rappresentare la punta di un nuovo *welfare state* in Italia, posto al centro di una rivoluzione del mondo del lavoro, la cui approvazione fu celebrata come abolizione della povertà, l'ultimo rapporto trimestrale Istat-VELA, pubblicato nel febbraio 2023, ha rappresentato come, al 31 dicembre 2022, il tasso di posti vacanti fosse pari al 2,3 per cento del totale dei disoccupati. quasi il massimo storico da quando, nel 2010, sono iniziate le rilevazioni di questo dato. Da anni, comunque, tale dato è in costante crescita, pur in presenza di un tasso di disoccupazione pari all'8,3 Da quando è stato introdotto il reddito di cittadinanza, ovvero in particolare nel 2019, il tasso dei posti vacanti non solo è aumentato, ma l'aumento è avvenuto con la massima velocità, passando in due anni da 1,4 a 2,3 per cento: vale a dire circa 200.000 posti vacanti in più, a dimostrazione del fatto che la misura in esame è un in esame è un deterrente al lavoro. L'inefficienza è aggravata anche dalle carenze dei sistemi informativi dei centri per l'impiego, che nei primi tre anni di applicazione della misura non si è inteso in alcun modo potenziare: cento dei centri per l'impiego dichiara di non avere una dotazione informatica in grado di dialogare con il sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), il 70 per cento con i sistemi informativi territoriali, cento non ha un sistema interoperabile con l'INPS e solo il 44 per cento dialoga con il sistema informativo unitario delle politiche per il lavoro (SIUPL); in questo contesto le informazioni non circolano tra gli attori a vario titolo coinvolti. Il Governo in carica sta affrontando gli effetti di queste politiche che si sono rivelate estremamente gravose quanto all'impatto sulla finanza pubblica, ma soprattutto totalmente inefficaci sul piano delle politiche attive, avendo generato, peraltro, effetti distorsivi nel mondo del lavoro le cui conseguenze investono in modo drammatico l'intero sistema produttivo. Tra queste conseguenze desta particolare preoccupazione la condizione di difficoltà per le imprese di reperire personale, soprattutto in possesso di competenze specifiche, che consenta di superare gli ostacoli

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro, con particolare riferimento alle novità previste in merito alle innovazioni tecnologiche, anche al fine di favorire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro e da Unioncamere, nel mese di maggio 2023 si è registrata una difficoltà di reperimento di risorse umane pari al 46,1 per cento, soprattutto a causa della mancanza dei candidati, con un aumento di circa otto punti percentuali rispetto alla media registrata nello stesso periodo del 2022, pur essendo circa 467.000 le assunzioni previste dalle imprese a maggio 2023 e oltre 1,5 milioni entro il mese di luglio. Al fine di incoraggiare e stimolare un più efficace incrocio tra domanda e offerta, il Governo ha previsto misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro declinate nel recente decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 attualmente in conversione. Nell'ambito di questo provvedimento si prevede all'articolo 5 l'istituzione del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa che sarà realizzato dall'INPS e gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito del predetto sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'assegno di inclusione e della misura per la formazione e il lavoro con l'obiettivo di agevolare la ricerca del lavoro, l'individuazione di attività di formazione, il rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili per la collettività, tenendo conto delle esperienze formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario nonché della disponibilità di di offerte di lavoro, corsi di formazione e ogni altro genere di intervento di politica attiva. La norma in questione nasce per superare alcune criticità connesse al reddito di cittadinanza e consentirà anche l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali esistenti per i soggetti accreditati al sistema sociale del lavoro, mettendo a fattor comune le informazioni informazioni sulle offerte di lavoro ed incrementando in tal modo la cooperazione tra pubblico e privato. La piattaforma inoltre garantirà anche le attività di monitoraggio, valutazione e controllo delle nuove misure di inclusione sociale ed attivazione al lavoro rispetto a cui si segnala anche il lavoro parallelo in corso di svolgimento di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche dei centri per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta già coordinando le attività con i diversi attori istituzionali chiamati a interagire nel complesso processo previsto dalle nuove misure. I lavori procedono in modo serrato e sono orientati a fornire nei tempi

il programma GOL destina gran parte delle sue risorse al finanziamento di percorsi di aggiornamento e di qualificazione dei beneficiari intercettati e accompagnati dai servizi verso un inserimento professionale. In questa prospettiva, il rafforzamento delle strutture tecnologiche e informatiche informatiche sopra richiamato si pone quale strumento utile per raggiungere queste finalità, rispetto a cui è necessaria la collaborazione di tutti gli attori della rete dei servizi per il lavoro. *(Applausi)*.

Ministro, colleghi, sottopongo oggi all'attenzione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che ringrazio per la sua disponibilità, una questione che riguarda le infrastrutture della Regione Marche e della città di Ancona: il raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara. È un'infrastruttura centrale, un'opera che sarà un volano per l'economia di tutta la Regione, in particolare per la città di Ancona, che ha delle straordinarie potenzialità. Città di mare che guarda ai Balcani, grazie al suo porto che occupa più di 6.500 lavoratori e genera il 3 per cento di tutto il PIL regionale, Ancona è geograficamente al centro dell'Italia e ha tutte le carte in regola per diventare un *hub* strategico del Sud Europa grazie a porto, aeroporto e interporto. Sono tre infrastrutture chiave che dialogano fra di loro e il loro sviluppo integrato è determinante per la crescita di Ancona, delle Marche e di tutto il Centro Italia. Se fino a quindici, vent'anni fa il cuore produttivo era formato dai distretti industriali di imprenditori come Francesco Merloni o Gennaro Pieralisi, oggi l'*asset* economico di questa area passa attraverso gli investimenti sui collegamenti e sulle sinergie infrastrutturali. La linea Orte-Falconara, che arriva ad Ancona passando dall'interporto di Jesi e arrivando all'aeroporto di Falconara, si inserisce in questo contesto. Proprio su questi temi (porto, aeroporto e interporto) ci sono già la massima attenzione e l'impegno tangibile del centrodestra al governo, che grazie a lei, signor Ministro, e al contributo importante del presidente della Regione Acquaroli, sta dando risposte concrete ai marchigiani: penso ai 20 milioni di fondi per l'aeroporto di Ancona e i suoi collegamenti con Milano, Roma e Napoli; ai 43 milioni per l'interporto delle Marche e, ancora, alle risorse del PNRR per il porto di Ancona. Il raddoppio della Orte-Falconara mira a rafforzare e velocizzare il collegamento tra i versanti Adriatico Adriatico e Tirrenico. Ancona e le Marche hanno straordinarie potenzialità. Per metterle a frutto bisogna lasciarsi alle spalle la politica dei «no» e, al contrario, aprire cantieri, realizzare opere, creare lavoro e futuro per questo territorio, come il centrodestra al Governo e lei, caro Ministro, state facendo. Ecco perché oggi le chiedo di indicare quali siano i tempi di realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, opera infrastrutturale strategica e necessaria per lo sviluppo economico di Ancona, delle Marche e di tutto il Centro Italia.

dopo nostra richiesta e vista la situazione in Emilia Romagna, hanno deciso di sospendere e rinviare a giugno lo sciopero del trasporto aereo che avevano fissato per

pur essendo sacro e legittimo il diritto di sciopero, in un momento drammatico come questo, non solo per i cittadini dell'Emilia Romagna e di parte delle Marche e della Toscana, rappresenti un bel segno di unità del Paese. Quindi, ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti. Arrivando alla questione del potenziamento e lo sviluppo dell'itinerario Orte-Falconara, è uno dei progetti ferroviari su cui abbiamo da subito, dal mese di ottobre, concentrato la nostra massima attenzione. È un intervento che, come diceva lei, si inserisce in un processo complessivo di potenziamento di tutta la rete. Entrando nel merito degli interventi previsti, su cui stiamo accelerando e correndo come matti, recuperando anche anche il tempo perduto in fase di ultimazione del PNRR, è in corso l'esecuzione dei seguenti lavori: raddoppio della tratta Spoleto-Campello, con previsione di attivazione entro la fine del 2024; nodo di Falconara per fasi successive, con la realizzazione della nuova stazione di Osimo (prima attivazione entro il 2026). È in fase di progettazione il raddoppio delle tratte Spoleto-Terni e Foligno-Fabriano e dei lotti 1 e 3 del raddoppio PM228-Castelplanio, con previsione di conclusione entro il corrente 2023. Abbiamo inoltre sbloccato gli *iter* approvativi per ulteriori due lotti finanziati con fondi PNRR, che saranno quindi doverosamente completati entro il 2026: il lotto PM228-Albacina e il lotto 2 Genga-Serra San Quirico. Con la conferenza dei servizi, chiusa lo scorso 26 aprile, entro il prossimo 26 maggio, è attesa la determinazione motivata da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici, del mio Ministero, con gara prevista entro il 15 giugno 2023. Infine, sempre con fondi PNRR, è prevista la velocizzazione di tratte prioritarie della Orte-Falconara. Grazie a tutte queste opere sarà possibile ridurre i tempi di percorrenza tra Roma e Ancona di oltre trenta minuti. Insomma, un processo sinergico di miglioramento per la crescita economica e sociale di cui potrà beneficiare l'intera Regione Marche. Capitolo a parte che affronterò - se vorremo - in un altro *question time* sono i lavori di messa in sicurezza della A14, su cui ho già fatto più di una riunione con i Governatori di Marche e Abruzzo e Autostrade per l'Italia.

una valutazione importante e positiva che l'impegno del Ministero sta dando per rendere protagonista la città di Ancona e le Marche nel caso specifico. Condivido con lei che la Orte-Falconara sia una tratta cruciale per lo sviluppo di tutto il territorio del Centro Italia. Credo che questA sia una delle

importanti nella rete ferroviaria, con continui cambi di orari, riduzione di treni, un servizio non all'altezza di un un posto così frequentato, mezzi sostitutivi non adeguati e persone obbligate ad attese lunghe in sottopassi improbabili. D'altra parte, oltre ai turisti, dobbiamo sempre pensare ai pendolari che utilizzano i treni per lavoro o per studio, e ovviamente hanno il diritto di avere un servizio funzionante. L'ultimo treno da Sestri Levante a La Spezia è alle 00:21, neanche un orario così *smart* per il turista che vuole rimanere, magari, di più alle Cinque Terre,

misure intenda adottare per aumentare il numero dei treni possibili e, in questa fase di manutenzione e di lavori, come ovviare a

Presidente, oggi la tratta ferroviaria Sestri Levante-La Spezia è servita da 55 collegamenti con treni regionali e regionali veloci durante i mesi invernali, offerta programmata sulla base delle richieste della Regione Liguria. Dalla metà di marzo alla prima domenica di novembre, in stagione turistica, si aggiungono i Cinque Terre Express, che servono la tratta Levanto-La Spezia per un totale di 99 treni regionali, al servizio sia dei pendolari che dei tanti turisti che visitano il parco delle Cinque Terre. Peraltro questi treni sono gli ultimissima generazione e offrono ben 611 posti a sedere, oltre al Inoltre, dallo scorso mese di aprile fino al 24 settembre si aggiungono i cosiddetti treni del mare, con altri quattro collegamenti tra La Spezia, Milano e Como nei fine settimana. Vorrei evidenziare che, sia nella stazione di La Spezia centrale che in tutte le località delle Cinque Terre, FS Security aumenterà il proprio personale per garantire la massima sicurezza di cittadini e turisti. Inoltre, stiamo già lavorando con Trenitalia per potenziare i collegamenti in vista del maggiore afflusso turistico previsto per l'estate. In particolare, in occasione dell'entrata in vigore dell'orario estivo di Trenitalia, sulle percorrenze *intercity* abbiamo già previsto modifiche alla programmazione per il rafforzamento dei collegamenti con la Liguria, sia per la riviera di Levante che per quella inoltre previsto un tavolo tecnico (a cui ovviamente le componenti parlamentari, a partire da voi che avete avuto il garbo di presentare questa interrogazione, sono da me previamente invitate) tra Trenitalia e Regione Liguria,

le esigenze di mobilità non riguardano solo le ferrovie, ma anche le strade (su cui stiamo lavorando), comprese le autostrade, e il trasporto aereo. Intendo quindi convocare nei prossimi giorni (e sicuramente prima dell'estate) una riunione con tutti i soggetti coinvolti, in modo da individuare soluzioni condivise in vista della prossima stagione estiva. ringrazio i colleghi per l'applauso che ci hanno rivolto, perché abbiamo posto una questione sacrosanta. In effetti, sarebbe auspicabile una risposta corale dei due Ministri che sono oggi coinvolti. Io apprezzo lo spirito della risposta del ministro Salvini, cioè il coinvolgimento anche dei parlamentari e delle istanze locali nel poter suggerire alcuni interventi. Questo è senz'altro un fatto buono e innovativo e voglio riconoscerlo. Il punto, però, è fatto di due questioni: la prima è che le Cinque Terre hanno avuto un'espansione enorme dal punto di vista turistico, sono

seconda questione. Noi siamo molto contenti dei turisti, però c'è un problema anche per i pendolari, per chi lavora; mi riferisco alla necessità di avere un treno di rientro per chi va a fare il cameriere, per chi va a lavare i piatti, per chi va a fare il bagnino e che però magari di sera si deve fermare a fare altre attività.

loro. Per questo le chiediamo, signor Ministro, non di aspettare la fine dell'estate o il tavolo, ma di chiedere che ci sia un treno che possa far rientrare questi lavoratori volenterosi nelle loro abitazioni subito dopo aver lavato i piatti, servito ai tavoli, eccetera. Questo vale ovviamente per le Cinque Terre, ma vale in assoluto in ogni parte del Paese dove ci sia uno sviluppo così ampio,

*question time* è diventata di strettissima attualità: un masso di grosse dimensioni è crollato ieri proprio sulla strada provinciale 562, denominata Mingardina, all'altezza del bivio della stazione di San Severo di Cento, una donna in auto è riuscita a frenare e si è salvata per miracolo. Proprio questa strada era stata riaperta dopo quasi cinque mesi di chiusura forzata a seguito dell'ordinanza sindacale del Comune di Camerota in provincia di Salerno. Con precedente ordinanza del dicembre 2022 emessa dal sindaco, veniva ordinata l'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili consistenti in un intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale su cui aggettano i versanti rocciosi pericolanti e prossimi al crollo. Quest'area rientra nel Piano paesaggistico del Cilento costiero, classificata come zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale. variando le modalità di demolizione delle formazioni ritenute instabili, si è dato luogo all'uso di esplosivi; successivamente, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e l'ente Parco nazionale del Cilento chiedevano al Comune di Camerota chiarimenti urgenti sui lavori. Con ordinanza del 27 marzo 2023 il sindaco di Camerota ha ordinato l'esecuzione sul tratto stradale compreso tra cala Finocchiara e spiaggia La Vela di lavori urgenti ed indifferibili finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza dello stesso tratto stradale e alla sua immediata riapertura. Con ordinanza del 30 marzo la Soprintendenza di Salerno ha disposto l'immediata sospensione delle attività previste nell'ordinanza sindacale citata del 27 marzo, salvo quanto strettamente necessario e indifferibile per scongiurare i pericoli derivanti dall'intervento *in itinere.* La strada provinciale 562 è stata riaperta a corsie alternate da semaforo mobile. Il 27 aprile è stato indetto un incontro a Salerno tra gli enti preposti e l'amministrazione comunale per tentare un accordo per il ripristino dello stato dei luoghi. Voglio ricordare che la strada costituisce l'accesso principale a Marina di Camerota ed è utilizzata dai residenti per raggiungere gli ospedali e i plessi scolastici superiori di Vallo della Lucania e Sapri,

e sono sempre più convinto del fatto che la reintroduzione di Province vere, elette direttamente dai cittadini, con poteri, denari e competenze, possa questo perché in questa sede io posso solo riferire quello che altri enti protagonisti mi hanno detto di una strada che rientra nella gestione della Provincia di Salerno inserita sia all'interno del Parco nazionale del Cilento che della zona speciale di conservazione Scoglio del Mingardo e gli ostacoli di natura amministrativa sono di competenza prevalente del Ministero della cultura. Io posso pertanto riferire - e lo faccio volentieri - quello che i Ministeri dell'interno, della cultura e dell'ambiente mi hanno predisposto. La mia considerazione, a monte, è che se la strada è statale - stamattina ho incontrato gli amministratori lucani che si occupano di Maratea, dove c'è stata una frana - interviene Anas, ne rispondo io ed entro il 15 luglio la strada va riaperta. In questo caso, io posso sollecitare, stimolare e agevolare. La prefettura ha invitato a procedere celermente alla messa in sicurezza del costone. Il sindaco del Comune di Camerota ha adottato diverse ordinanze per l'esecuzione di lavori indifferibili e urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata Tuttavia, nello scorso mese di marzo, sia l'ente Parco nazionale del Cilento, sia la Soprintendenza archeologica delle Province di Salerno e Avellino hanno disposto l'immediata sospensione dei lavori in quanto l'amministrazione comunale non aveva richiesto il nulla osta e le autorizzazioni necessarie. Sia la Soprintendenza che l'ente parco hanno ribadito di ritenere ammissibili, al fine di consentire l'eliminazione dell'imminente pericolo, i soli interventi volti alla rimozione chirurgica dei massi in imminente pericolo di crollo, con connessa pulizia della carreggiata dal materiale. Poi servirà un vocabolario per tradurre dal linguaggio della Soprintendenza a quello del comune cittadino che cosa ciò va a significare. Indi il sindaco del Comune di Camerota ha avviato i lavori di rimozione di un ammasso roccioso sulla carreggiata e lo scorso 20 aprile ha disposto la riapertura temporanea e parziale a senso unico alternato del traffico veicolare. Il 12 maggio scorso la Soprintendenza ha scritto al Comune di Camerota una nota con la quale ha ribadito che, per gli interventi che rivestono carattere di urgenza, la disciplina paesaggistica non contempla deroghe e quindi il Comune dovrà conseguire e attivare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Al contempo, ha ribadito la propria disponibilità a rendere il parere di competenza con la massima urgenza. Auspico che - questo posso fare per serietà sulla base di questa disponibilità da parte tutti gli enti coinvolti, si possa giungere a una rapida risoluzione della vicenda, per garantire - questo ci interessa - la riapertura totale e in sicurezza della Mingardina, anche in considerazione dell'imminente avvio della stagione estiva. Quindi, tradotto, posso chiamare il sindaco, il Presidente della Provincia, l'ente parco e il soprintendente, chiedendo loro di mettersi d'accordo e di fare in fretta. Ministro, la ringrazio. Sono convinto che l'interrogazione vada in questo senso e che lei sia la persona giusta per risolvere questo problema, perché se non si mettono d'accordo gli enti coinvolti, le conseguenze vanno a scapito dei cittadini. La ringrazio per il suo interessamento e sono soddisfatto.

la vicinanza agli alluvionati e il cordoglio alle famiglie delle vittime. Signor Ministro, gli investimenti in opere pubbliche portano benefici concreti a tutta la collettività. Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità di merci e di persone efficace ed efficiente, che possa sostenere la crescita sostenibile a lungo termine di un territorio, oltre che incrementarne l'attrattività e consolidarne le capacità competitive. In Sicilia sono presenti circa 140 opere infrastrutturali incompiute o il cui termine contrattuale per l'ultimazione è già superato. Si tratta di oltre il 30 per cento del dato complessivo nazionale e di un dispendio di risorse che supererebbe i 400 milioni di euro: strade e autostrade, ma anche opere idriche e porti, che rappresentano un'enorme occasione di sviluppo per la nostra bella Regione. C'è poi l'annoso problema delle reti ferroviarie siciliane. Infatti le località servite sono 173, con 1.369 chilometri di linea ferrata, di cui soltanto 791 sono elettrificati, e con un doppio binario soltanto per 223 chilometri, mentre abbiamo ancora 568 chilometri a binario unico. Il ponte sullo Stretto di Messina, oltre a essere un'opera strategica per l'Italia, in grado di contribuire alla riduzione del divario Nord-Sud, lo è anche per l'Europa, con l'obiettivo di completare il corridoio scandinavo-mediterraneo delle reti transeuropee di trasporto TEN-T, e costituisce anche uno snodo fondamentale per la velocizzazione delle nostre ferrovie. Sono altrettanto urgenti e necessari gli interventi finalizzati a un miglioramento complessivo delle reti viarie e autostradali della Regione, anche connesse al ponte sullo Stretto, nonché finalizzati alla realizzazione di tutte le infrastrutture di supporto fondamentali per riuscire a sfruttare appieno tutte le potenzialità dell'opera e metterle al servizio della Sicilia, del Mezzogiorno e dell'Italia. Vorrei sapere quindi, signor Ministro, quali iniziative di competenza intenda adottare per realizzare un piano di investimenti in infrastrutture efficienti e strategiche per la Regione Sicilia.

come rete di connessione Nord-Sud da ultimare entro il 2030. Probabilmente non ci arriveremo per il 2030, però sicuramente non andremo molto oltre. Se lei mi avesse interrogato qualche anno fa, la risposta sarebbe stata diversa, perché solo il ponte non risolve i problemi di nessuno; il ponte, inserito in un contesto che in questi due minuti a mia disposizione vado a riassumere, ha assolutamente un senso diverso. Nel decreto-legge ponte, infatti, abbiamo previsto ad esempio per il completamento della A19 Palermo-Catania la nomina di un commissario straordinario per superare quelle lunghezze. Vi sono interventi programmati in Sicilia altrettanti sono in corso in Calabria. Per la sola rete stradale nazionale sono programmati investimenti per circa 15 miliardi di euro. Cito ad esempio la Ragusa-Catania (un investimento di 1,5 miliardi di euro), per i cui lavori sarò in visita la settimana prossima; l'adeguamento a quattro corsie della strada statale 640, la "Strada degli scrittori" (Agrigento-Caltanissetta), con un investimento di 1 miliardo di euro; il raddoppio della carreggiata sulla strada statale 284 tra Paternò e Adrano 500 milioni di euro. È in corso di aggiudicazione la tangenziale di Gela, per un investimento di 400 milioni di euro. Potrei andare avanti, ma vi annoierei. Sono in corso le attività di progettazione della tangenziale di Palermo, della tangenziale di Agrigento, della tangenziale di Catania e del collegamento Trapani-Mazara del Vallo-Marsala. Per il settore autostradale sono in corso il nono lotto dell'autostrada Siracusa-Gela, per un investimento di 500 milioni di euro e la riqualificazione della A18, della A19 e della A20, per altri 100 milioni di euro. Passando alla rete ferroviaria, in Sicilia sono già programmati investimenti per circa 13 miliardi di euro. Per il nuovo collegamento Palermo-Catania-Messina è previsto un investimento coperto di 11,2 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di realizzare 148 chilometri di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci, entro giugno 2026. Cito inoltre il ripristino e l'elettrificazione della Palermo-Trapani via Milo, per altri 280 milioni di euro; il *bypass* di Augusta, per 172 milioni di euro. Prevediamo anche interventi per il nodo di Palermo e il nodo di Catania, per la linea Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, per il collegamento con gli aeroporti di Trapani e di Fontanarossa, per la Caltagirone-Gela, con un investimento complessivo di altri 600 milioni di euro. Riassumendo, il ponte da solo non risolve i problemi di nessuno; il ponte, inserito come pezzo di un *puzzle* che prevede decine di miliardi di investimenti tra Sicilia e Calabria, è un'opera necessaria di cui l'Italia andrà orgogliosa per il mondo.

purtroppo, avendo visto passare tanti Governi, tanti Ministri, tante passerelle, sono comprensibilmente sfiduciati. La sfiducia viene dal fatto che negli anni tanti siciliani sono stati chiamati a ricoprire ruoli importanti nei palazzi romani, ma purtroppo i risultati non sono stati quelli sperati. La Sicilia è cresciuta: sì, è vero, è cresciuta, ma io dico che è una crescita naturale fisiologica e non è stata certamente purtroppo una crescita sostenuta da quei siciliani che a Roma hanno ricoperto incarichi importanti in occasioni irripetibili.

che un Ministro dei lavori pubblici così attivo, così operativo e così attento alle problematiche del Mezzogiorno davvero non l'abbiamo mai visto, forse non l'abbiamo mai avuto. Per giunta, non è un Ministro siciliano, ma un Ministro milanese. Un motivo di tutta questa grande attenzione al Sud c'è: perché è un grande *leader* di partito, che non è più quel partito che difendeva soltanto le ragioni di una parte del Paese; oggi la Lega è un partito nazionale che, grazie alla sua lungimirante visione, sa bene che non può esserci un'Italia a due velocità. Qui interviene la sua quasi ossessione per la realizzazione del ponte sullo Stretto, giustamente, ricordando il provvedimento che abbiamo incardinato ieri in Commissione di cui mi onoro di essere anche relatore. Lei, Ministro, come tanti siciliani onesti e lavoratori che credono in una Sicilia migliore e che oggi stanno riacquistando fiducia grazie anche al suo incessante lavoro, ha ben compreso che il ponte è l'unica - dico anche ultima - opportunità per il Sud per recuperare quel *gap* infrastrutturale che ci divide dal resto del Paese. La ringrazio pertanto a nome mio e di tanti siciliani e mi complimento per il lavoro che sta svolgendo. Con lo *slogan* che ho fatto mio, "Ponte e libertà", mi dichiaro ampiamente soddisfatto.

*(PD-IDP)*. Ministro Salvini, mi rivolgo a lei oggi per affrontare una questione di grande importanza per il principale scalo commerciale del Paese, il porto di Genova. Come lei ben sa, sono stati pianificati e impegnati ingenti investimenti per il suo sviluppo e per le relative infrastrutture di collegamento. Parliamo di miliardi di euro di risorse pubbliche destinati alla costruzione della nuova diga, al Terzo Valico dei Giovi, alla gronda autostradale e ad altre opere infrastrutturali al servizio del porto e della città. Tuttavia, molte problematiche si stanno affacciando su queste opere a causa di una pessima gestione che sta mettendo a rischio i tempi di realizzazione e le ricadute positive sulla città e sui suoi abitanti. Emblematico è il tema che le sottopongo oggi della riconosciuta esigenza di spostare i depositi chimici costieri di Carmagnani e Superba dalla zona di Genova Multedo, una richiesta che proviene dalla popolazione residente, che ha evidenziato da tempo problemi di vivibilità e sicurezza, preoccupazioni che ribadiscono giustamente anche i cittadini genovesi che vivono a poca distanza dal luogo che il sindaco ha scelto per il dislocamento. L'ubicazione proposta presenta, infatti, gravi problemi ambientali, sociali e occupazionali. I materiali che sarebbero stoccati e movimentati a Sampierdarena sono infatti infiammabili, tossici e pericolosi per l'ambiente, come indicato nella documentazione ufficiale e sarebbero collocati a soli 300 metri dalle abitazioni, in uno dei quartieri più densamente abitati della città. Si prevede che, oltre a diversi treni, 30 autobotti al giorno trasportino tali materiali pericolosi per le strade cittadine. Va inoltre considerato che è vigente un'ordinanza della Capitaneria di porto che vieta l'ormeggio e il transito di navi cisterna di prodotti petroliferi e petrolchimici

regolatore portuale per destinare aree attualmente utilizzate per il traffico merci a scopo di deposito di sostanze chimiche? Non ritiene opportuno, considerata l'ingente cifra di 30 milioni di euro di risorse pubbliche destinate al progetto di ricollocazione, che tali risorse siano utilizzate, non per ampliare depositi, ma in modo più efficace per trovare una soluzione urbanistica che consenta di trasferire le attività dei depositi in un'area distante dalle abitazioni e che non comprometta il traffico merci attuale e l'occupazione nel porto di Genova? Le chiedo, signor Ministro, di fornire risposte a queste domande cruciali per il futuro del principale porto italiano,

Ringrazio per l'interrogazione. È vero, Genova vive e vivrà uno sviluppo straordinario con il combinato disposto di diga, *waterfront*, porto, terzo valico e logistica ad Alessandria: tutto ciò permetterà al triangolo industriale Genova-Torino-Milano di tornare a essere la perla che era. Posso rispondere - e lo faccio nel dettaglio come i senatori interroganti giustamente meritano - su scelte che io ho trovato sulla scrivania, fatte da Ministri che mi hanno preceduto. La delocalizzazione dei depositi per prodotti chimici di Multedo è infatti un tema affrontato da diversi anni, sia dai gestori degli stessi depositi che dall'amministrazione comunale, in quanto l'attuale localizzazione presenta una critica convivenza, come ricordato, con il contesto urbano residenziale. Sul tema l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha riferito che la ridislocazione dei depositi costieri è un progetto inserito nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e, quindi, non può comportare - a giudizio dell'Autorità portuale stessa - perdite di traffico merci e di occupazione. Infatti, la ricollocazione deve tener conto dell'obiettivo prioritario del complessivo mantenimento dei livelli occupazionali, dei traffici e dello sviluppo degli investimenti. Veniamo ai tempi. Con le modifiche apportate al piano regolatore portuale, l'adeguamento tecnico-funzionale ha previsto l'individuazione dell'area di Sampierdarena, adottata con delibera del Comitato di gestione del 15 dicembre 2021, sulla quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole a settembre 2022. Quanto all'impatto sulla rete ferroviaria, abbiamo approfondito che non si rilevano conseguenze significative, in quanto mera ricollocazione di attività già insediate nel territorio genovese. Aggiungo che in ambito portuale sono in atto rilevanti investimenti di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, che prevedono anche la realizzazione di interventi dedicati specificamente alle merci cosiddette pericolose e ciò in linea, peraltro, con le direttive comunitarie. Infine, evidenzio come la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti chimici costituiscano attività di interesse portuale da sempre sviluppate nello scalo di Genova, rientranti in quella multi funzionalità che caratterizza obiettivi contenuti del vigente piano regolatore portuale. Pertanto, la possibilità di rilocalizzare i depositi chimici al di fuori del contesto abitativo di Multedo è sempre stata posta nella logica di una migliore convivenza tra attività portuale e ambito urbano. ambito urbano. L'istruttoria dell'adeguamento tecnico funzionale, risalente al 2021, si è basata su analisi tecniche e studi ambientali che non hanno rilevato nessun aumento del carico ambientale. La delibera stessa del comitato di gestione del 30 dicembre 2021 ha previsto espressamente che il contributo di 30 milioni, cui lei faceva riferimento, debba essere destinato a garantire maggiore sicurezza, incremento della tutela ambientale ed il mantenimento di un'attività economica di rilevanza strategica.

questa scelta è una scelta che ha fatto e ha voluto il sindaco in carica, nonostante l'Autorità di sistema portuale avesse fatto uno studio che aveva analizzato la situazione e trovato soluzioni differenti. Non posso ritenermi soddisfatto perché, come le dicevo prima, c'è una perdita occupazionale. Questa è stata dichiarata dai sindacati, dagli imprenditori, dal principale armatore italiano, che dirà che lì disinvestirà Non posso ritenermi soddisfatto perché, se è giusto spostare, come lei giustamente ricordava e come io condivido, quei depositi chimici da un luogo vicino alle case, a una distanza di 50 metri dalle case, non per questo si possono spostare a 300 metri dalle case. Quei 30 milioni non vengono usati solo per la ricollocazione, ma per ampliare quei depositi

andrebbe a compromettere la sicurezza e la salute dei cittadini genovesi. *(Applausi)*.

Signor Presidente, signor Ministro, il fenomeno delle locazioni brevi turistiche sta impattando ormai da tempo negativamente sulla vivibilità di grandi città, delle città d'arte e di importanti località turistiche italiane, causando lo spopolamento dei residenti dai centri storici e trasformando il tessuto urbano, tra usi turistici e usi residenziali. Parlo di alcune importanti città come Venezia, Verona, Milano, Firenze e Roma, ma anche di piccole località turistiche che vantano milioni di presenze, come il mio paese, Malcesine, e come tutto il lago di Garda da cui provengo. La forte riduzione della disponibilità di alloggi per affitti a lungo termine e il caro affitti, con l'impennata dei canoni, aggravata dalla pressione della domanda turistica rende estremamente difficoltoso trovare alloggi economicamente accessibili nelle città e in diverse località turistiche: per i giovani studenti (pensiamo solo alla loro giusta protesta in tenda delle ultime settimane), ma anche per famiglie e lavoratori e per lo stesso personale del comparto turistico. situazione che aggravava la già persistente difficoltà di reperimento di personale da parte delle imprese turistiche. Lo spopolamento dei centri storici comporta, a livello turistico, una consistente perdita di attrattività, di autenticità e vivacità, di quella italianità tanto ricercata dai turisti. Non si può e non si deve inoltre trascurare la dimensione di un turismo sostenibile che tenga pienamente conto dei suoi impatti economici, sociali e ambientali attuali e futuri, rispondendo alle esigenze dei visitatori, dell'industria turistica, dell'ambiente e delle comunità ospitanti. Occorre quindi trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di disciplinare gli affitti brevi, la tutela del diritto alla residenza e il diritto di svolgere l'attività di locazione turistica. Urge la necessità di una regolamentazione omogenea e uniforme a livello nazionale che tenga conto delle tipicità dei diversi territori e della prospettiva abitativa e urbanistica per proteggere il tessuto residenziale e socioeconomico dei quartieri. Considerato quanto sopra, si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro per trovare una soluzione concreta che regolamenti il fenomeno relativo alle locazioni brevi di tipo turistico, ormai fuori controllo, e per rispondere parallelamente all'esigenza di favorire il ripopolamento dei centri storici.

che mi offre la possibilità di spiegare quali sono le intenzioni e le proposte che a breve farà il Ministero, avendo ascoltato tutte le associazioni di categoria, i sindaci i sindaci delle città metropolitane e i sindacati dei condomini. Il fenomeno degli affitti brevi, come lei sa, è ampiamente diffuso in Europa; non nasce oggi,

Per quanto riguarda la finalità turistica, tali locazioni hanno di certo contribuito alla ripresa di flussi turistici in Italia, generando ricadute in termini di turismo che a volte, come ha detto lei, è sovradimensionato, così come in termini di vivibilità dei centri urbani, a causa del frequente *turnover* turistico che impatta spesso negativamente sulla qualità e sulla vita dei residenti. Queste ed altre problematiche legate al fenomeno sono al centro del tavolo di lavoro istituito recentemente presso il mio Dicastero insieme agli amministratori locali e alle principali associazioni di categoria per per far chiarezza sull'attuale assetto normativo delle locazioni turistiche, ad oggi caratterizzato principalmente a livello regionale con regolamenti comunali molto spesso disomogenei. L'obiettivo comune è quello di delineare una cornice normativa da applicare sul territorio nazionale che tenga conto del divario esistente ad oggi tra i vari Comuni italiani in termini di densità turistica e capacità ricettiva. Un ultimo incontro al tavolo tecnico si è tenuto proprio con l'associazione degli inquilini. Alla luce di tali lavori e prendendo in considerazione le proposte formulate dagli *stakeholder*, gli uffici del Ministero del turismo stanno predisponendo un disegno di legge volto a definire la locazione per finalità turistiche e a fissarne limiti e condizioni anche qualora svolta in forma imprenditoriale. La legge prevederà in particolare apposite sanzioni volte a contrastare forme irregolari di ospitalità e a garantire la tutela della concorrenza e della sicurezza dei territori. Ciò avverrà soprattutto nella fase attuativa, in stretta sinergia con le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle competenze che contraddistinguono i livelli di governo. È mia intenzione pertanto tener fede all'impegno assunto introducendo una disciplina nazionale delle locazioni turistiche che rappresenti un punto di equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata e la tutela dei contesti e la tutela dei contesti socio-economici locali. la Ministra per la sua risposta, ma francamente non posso ritenermi soddisfatta. Mi aspettavo che entrasse più nel merito e nello specifico della proposta di legge

nel vago. Aspetteremo questa proposta per analizzarla e confrontarci sulla sua praticabilità in un secondo momento. Tengo a ribadire di nuovo l'importanza di dare sostegno anche ai Comuni piccoli, che vantano milioni di presenze turistiche, perché hanno bisogno di una normativa a carattere nazionale, perché con i regolamenti comunali non sono in grado, senza una condotta a livello nazionale, di operare sul territorio. Faccio presente che non si tratta di criminalizzare il fenomeno, che è esploso negli ultimi anni, delle locazioni brevi, ma d'altro canto abbiamo un settore alberghiero che è iper-regolamentato e quindi, giustamente, va regolamentato anche questo. Tramite questa regolamentazione si lavorerà anche Le chiedo particolare attenzione anche per quanto riguarda una revisione a trecentosessanta gradi degli affitti in genere, perché dobbiamo anche tutelare il diritto alla residenza e agli affitti a lungo termine, creando una rete di protezione che tuteli sia i proprietari, sia

- Premesso che: i dati sui primi mesi del 2023 confermano le previsioni che individuano nel 2023 l'anno determinante per sancire il ritorno delle presenze turistiche a livelli precedenti al 2020, dopo le pesantissime perdite provocate dalla pandemia; secondo i dati di "Demoskopica", si stimano 127 milioni di arrivi, con un rialzo dell'11,2 per cento sul 2022 e un conseguente incremento consistente della domanda di lavoro; si assiste però al paradosso per il quale alle maggiori opportunità di lavoro si contrappone l'allarme lanciato dagli operatori del settore

Secondo i dati forniti da Assoturismo e Confesercenti, mancano i profili più ricercati, come addetti specializzati e professioni non qualificate. La difficoltà nel reperire personale nel settore turistico, in particolare nei settori del comparto caratterizzati da un'elevata stagionalità, ha ormai assunto dimensioni strutturali e si è manifestata regolarmente anche negli anni precedenti all'emergenza pandemica, ma la ricerca di una soluzione duratura diventa di massima urgenza in questo momento, che è cruciale per la ripartenza del comparto. Il 15 marzo scorso si è tenuto il primo incontro del tavolo di lavoro tra Ministero del turismo e associazioni di categoria. Considerato che lei, Ministro, ha trasmesso alle Camere il Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027, nel quale, a margine di una serie di buoni e condivisibili propositi, non si intravedono risposte concrete alle citate criticità, l'unica risposta che ad oggi il Governo sembra aver voluto dare è il ritorno a forme contrattuali che precarizzano ulteriormente il lavoro e che riducono i diritti e le tutele dei lavoratori con il ritorno dei cosiddetti *voucher*, il cui utilizzo è stato addirittura ampliato con l'ultimo decreto lavoro per il settore termale, delle fiere e dei parchi divertimento. Non si hanno notizie, invece, della pur annunciata sospensione del limite dei ventinove anni per l'apprendistato professionalizzante. Per le imprese che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari è possibile stimare una perdita media di fatturato intorno al 5,3 con il rischio di un conseguente abbassamento degli *standard* qualitativi. Si chiede di sapere quali iniziative lei, Ministra, intenda adottare con la massima urgenza per dare una risposta concreta alle imprese che vedono compromesso il proprio potenziale produttivo in un momento così determinante per la ripresa del comparto; se non ritenga opportuno intervenire con un provvedimento *ad hoc* per il settore turistico, contenente le strategie necessarie a garantire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso una pianificazione efficace delle politiche attive del lavoro,

la carenza di personale nel comparto turistico, specialmente stagionale, rappresenta certamente una criticità, che rischia di ridurre l'impatto positivo della ripresa del settore. Per risolverlo bisogna garantire maggiore flessibilità contrattuale e rafforzare politiche attive per la formazione. A tal proposito, ho dato incarico ai miei uffici di elaborare un pacchetto di norme dedicate sia ai lavoratori che ai datori di lavoro del comparto turistico. Nello specifico, la finalità delle disposizioni in questione è, da una parte, quella di agevolare le imprese del settore per quanto riguarda l'assunzione di nuovo personale; dall'altra, di indurre i lavoratori a presentare candidature per svolgere la propria attività lavorativa in ambito turistico. A titolo di esempio, un primo intervento è stato rivolto al contratto di formazione lavoro per il turismo, che consentirebbe alle associazioni e alle imprese del comparto turistico alberghiero sottolineare strutturale - difficoltà di reperimento di personale da parte delle imprese operanti nel settore, agevolando notevolmente l'occupazione giovanile e garantendo l'acquisizione di una qualificazione di alto livello derivante dalla formazione *on the job*, e in generale la ripresa e il rilancio dell'intero comparto. Tra le misure che stiamo esaminando vi è poi quella relativa all'esonero contributivo a favore dei lavoratori del turismo, che consentirebbe ai datori di lavoro privati nel settore turistico di essere esonerati dai contributi previdenziali, e quella concernente la tassazione agevolata dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo in età pensionabile o in quiescenza diretta; quindi, consentirebbe di incentivare il mantenimento in servizio dei lavoratori già in possesso di requisiti pensionistici, che permetterebbe di fare emergere un'importante fetta di lavoro sommerso e anche di non disperdere quello che è un patrimonio di professionalità e di competenze utili anche per formare i giovani. Al fine di consentire l'assunzione di persone - come ha chiesto lei - di età superiore a ventinove anni nel settore turistico alberghiero, è allo studio una norma disciplinante l'apprendistato professionalizzante per il settore turistico, che costituirebbe un valido strumento per aumentare il numero di lavoratori nel settore turistico, allo stesso tempo offrendo loro un'alta qualificazione professionale. Inoltre, per sopperire alla strutturale difficoltà di reperimento del personale impiegato per attività di lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero, ivi compreso quello termale, si è pensato di introdurre misure di semplificazione delle procedure di assunzione di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea, già in possesso di visto di ingresso o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi da quelli lavorativi. Per l'attuazione di tali interventi il mio Dicastero sta già lavorando con il Ministero del lavoro dando avvio a una proficua interlocuzione, proprio al fine di intervenire in modo tempestivo sul problema della mancanza di personale. A tal proposito, in data a 15 marzo 2023, si è tenuto un primo incontro tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, nel corso del quale peraltro è emersa la necessità di rivolgersi in particolare alle nuove generazioni, raccontando loro

ringrazio la signora Ministro ma non posso ritenermi soddisfatto dalle sue risposte. I ritardi fin qui accumulati di sicuro avranno già compromesso la stagione 2023. Mi permetta poi di porre in evidenza il fatto che l'utilizzo delle prestazioni occasionali è assolutamente inadeguato a far emergere il lavoro sommerso, mentre al contrario diventa uno strumento di agevolazione di forme di lavoro irregolari. Negli anni in cui si è fatto ricorso ai *voucher,* solo il 20 per cento di questi era riferito al settore turistico ed ora, a pochi mesi dalla loro reintroduzione, l'ispezione svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro ha riscontrato irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest: su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori in nero, fra cui 16 minori e 101 lavoratori extracomunitari, tra i quali 18 senza permessi di soggiorno. Si auspica quindi che lei voglia impegnarsi per assicurare il tempestivo e capillare controllo delle situazioni di irregolarità. Ribadiamo la necessità di affrontare il problema in un'ottica di sistema, attraverso un provvedimento *ad hoc,* per risolvere in modo strutturale la carenza di personale e trovare soluzioni efficaci per garantire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, visto che, anche laddove esistono strumenti contrattuali vantaggiosi per il lavoratore (vedi quello del bagnino di salvataggio), permane una strutturale carenza di personale.

Grazie a tutte Grazie